«Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021» La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche al calendario corrente e il calendario dei lavori fino al 24 marzo. In relazione all'*iter* in Commissione del decreto-legge sul funzionamento del CONI, la discussione del provvedimento avrà inizio domani alle ore 10, per proseguire, ove non conclusa, nella giornata di martedì 16 marzo alle ore 16,30. Le settimane dal 15 al 19 e dal 22 al 26 marzo saranno prevalentemente riservate ai lavori delle Commissioni. L'Assemblea si riunirà inoltre mercoledì 24 marzo, alle ore 9, per le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 25 e 26 marzo

Questa è la mia opinione. Quando lei prenderà la parola, dirà la sua. Tornando al tema, il *cashback* è materia di enorme attualità, perché - se non sbaglio - la settimana prossima il Consiglio dei ministri dovrà finalmente

una mozione che riguarda la sospensione del *cashback* potrebbe essere utile a tutti in quest'ottica. Qual è lo scopo della mozione? Il ricavato - stiamo parlando di quasi 5 miliardi di euro - potrebbe essere

inutilmente esosa e poco efficace. Non è il tempo dei premi, delle riffe. Non è il tempo di questo tipo di misure. Servono aiuti concreti ed è per questo che nella mozione Fratelli d'Italia chiede la sospensione del *cashback* e l'investimento delle risorse ricavate - ripeto, quasi 5 miliardi di euro - per indennizzare i settori colpiti. Mi pare strano che, di fronte a questa proposta, ci sia la totale insensibilità da parte della maggioranza.

il parere sul *recovery plan*, ma noi non abbiamo ancora capito se è lo stesso del Governo precedente o se c'è una nuova versione.

Alla luce di tutte queste problematiche - *recovery plan* del Governo precedente, quello del Governo attuale e cosa deve fare il Parlamento

dell'opposizione. Per questo motivo, e non per altro, voteremo contro la proposta di modifica del calendario

come ipotizzare che essa sia subordinata a seconda che il *recovery plan* dica una cosa piuttosto che un'altra. Non possiamo, però, accedere alla tesi

del Governo - noi, forza di opposizione, dobbiamo rimanere passivamente in attesa che il Senato esprima una decisione su una nostra mozione che - come tutti sanno - è diversa da una legge cogente. Pertanto, riconfermiamo la richiesta ai colleghi di accedere alla proposta formulata dalla senatrice Rauti e di votare a favore della modifica del calendario dei

favore nei confronti della proposta e del suo contenuto.

nel calendario la mozione sul *cashback*.

Toni Comin e Clara Ponsati. È solo l'ultima puntata di una questione che è nuovamente esplosa nel 2010 quando il tribunale costituzionale di Madrid ha riscritto 14 articoli dello Statuto di autonomia, in vigore dal 2006, minandone l'impianto autonomistico di autogoverno. Dopo quella decisione, il Governo di Madrid non ha voluto più riaprire un confronto ed è su quelle basi che hanno trovato nuovo alimento le spinte separatiste che hanno avuto il loro culmine nel *referendum* dell'autunno del 2017. Nei giorni che lo precedettero, come autonomisti, la scorsa legislatura presentammo un'interpellanza urgente per chiedere all'Italia di farsi promotrice di dialogo. Oggi, come allora, crediamo che l'Europa debba aiutare il percorso per il riconoscimento di forme più ampie di autogoverno rispettose della storia e della specificità catalana e in grado di rimarginare le profonde ferite del rapporto tra questa importante Regione e l'autorità centrale. È proprio nelle situazioni di crisi che i principi fondativi devono far valere il loro peso, quelli di Ventotene e della dichiarazione di Chivasso, per un'Europa federale dei popoli e delle regioni. Non sono un vezzo, ma solo premessa e condizione per una sempre maggior solidarietà e dialogo come strada per la risoluzione di tutti i conflitti. Il nostro Gruppo Per le Autonomie esprime solidarietà alla Catalogna, ai suoi eurodeputati e a tutti quei popoli che hanno il diritto di vivere secondo la propria cultura, le proprie tradizioni e la propria lingua.

Signor Presidente, rom significa uomo libero e i rom portano nel sangue l'indole della loro libertà culturale e sociale. È perciò impensabile chiedere di tradire le proprie identità rinunciando a vivere in maniera diversa dalle loro tradizioni. Chiedere la carità anziché lavorare fa parte del loro essere ed è impensabile negarglielo e, se l'Europa indica l'Italia come la Nazione con la minor percentuale di presenza rom, a questo punto abbiamo un grosso problema perché - per fortuna sono pochi - non sappiamo né quanti, né dove sono. È perciò importante avere un vero monitoraggio e un censimento, visto che l'ultimo è inaffidabile e risale al 2008. Si deve rispettare la loro cultura, ma occorre prima far loro rispettare le leggi e la cultura italiana, perché non tutti giustificano che siano liberi e senza regole e poi alcuni girino in Ferrari o Lamborghini acquistate non si sa come. Libertà per i rom, ma rispetto per tutti, a cominciare dallo spendere bene i soldi per veri progetti di integrazione e convivenza, specialmente a Roma dove il sindaco Raggi, oltre a non rispettare i suoi cittadini, provoca quelli delle province del Lazio *(Applausi)*: un solo insediamento illegale chiuso e, a fronte della chiusura,

spinge i rom fuori Roma, senza interessarsi a dove e come ciò avvenga: non trova una meta se non a Frosinone, Rieti, Latina o Viterbo? Raggi vuole usare buchi di entrata delle altre province laziali, ma - come già per i rifiuti ed ora per i rom - ripeto al sindaco che Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo non sono né la pattumiera né tantomeno il campo rom di Roma. Le province amano Roma e sono pronte a condividere progetti e necessità, ma non a subirli, soprattutto con avvertimenti inopportuni *(Applausi)*. Roma ha bisogno di tornare ad essere Roma

Presidente, il Ministro della salute ha firmato l'ordinanza che proroga la sospensione dell'attività degli allevamenti di visoni in tutto il territorio italiano fino al 31 dicembre 2021. La decisione di prolungare la sospensione arriva dopo un primo stop a novembre e dopo un nuovo *report* dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare in cui si ribadiva il rischio di diffusione di varianti pericolose tra furetti e visoni. In questo modo non solo è stata riconosciuta l'efficacia e la necessità di detto intervento come ulteriore misura per combattere la diffusione del coronavirus e così tutelare la salute pubblica, ma è stata altresì risparmiata la vita a migliaia di cuccioli di animali - circa 35.000 in questo solo anno - sottraendoli a indicibili sofferenze causate dagli allevamenti intensivi. Infatti, i visoni degli allevamenti intensivi sono destinati a essere uccisi con il gas per diventare delle pellicce dopo otto o nove mesi di prigionia, costretti in minuscole gabbie di rete metallica. Attualmente sono sei gli allevamenti presenti in Italia, in alcuni dei quali sono stati abbattuti migliaia di visoni per bloccare proprio la diffusione del coronavirus, ma ci sono ancora molti focolai e il monitoraggio costerà alla sanità pubblica circa 250.000 euro in un anno. In considerazione della scarsa efficacia dello *screening* così come è stato, soprattutto per l'elevato rischio di ulteriore diffusione del virus anche in forma mutata, come provano le evidenze scientifiche, è necessario che l'allevamento dei visoni sia vietato. I motivi che impongono questa soluzione non risiedono unicamente nell'esigenza della salute pubblica e di farlo tagliando dei costi economici elevati, ma vi sono anche ragioni etiche, morali, di giustizia, che chiedono che si ponga fine a questa smisurata sofferenza per gli animali. Sono già numerosi i Paesi europei che hanno detto addio all'allevamento intensivo di questi animali: Svizzera, Austria, Regno Unito, Repubblica Ceca, Serbia, Norvegia, Olanda, Svezia, Danimarca; l'Ungheria invece ha vietato l'importazione di visoni come misura preventiva; la Francia li ha vietati a partire dal 2026. signor Presidente, auspico che questo Governo a guida Draghi e il ministro Speranza abbiano il coraggio di chiudere definitivamente questi allevamenti, aprire le gabbie e far vivere quei deliziosi e bellissimi animali quali sono i visoni. *(Applausi)*.

Signor Presidente, intervengo per porre all'attenzione dell'Assemblea la problematica sempre più presente nelle odierne pagine di cronaca, soprattutto in epoca Covid, dei soggetti affetti da patologie per le quali è necessaria l'assistenza domiciliare integrata. (ADI) è un insieme di servizi e interventi socio-sanitari erogati al paziente all'interno della sua abitazione. Avviene attraverso prestazioni da parte di diversi professionisti, con l'obiettivo di evitare, per quanto possibile, il ricovero del paziente in ospedale o la sua collocazione in una struttura residenziale oltre il tempo strettamente necessario. Si tratta di un servizio domiciliare in grado di evitare una situazione traumatica per il paziente, oltre che un aggravio dei costi per l'assistenza in termini economici. Tuttavia, le procedure e le tipologie assistenziali di ADI non sembrano essere soluzione sufficiente per tante famiglie italiane. Sono sempre più numerose le richieste d'aiuto, le grida di disperazione delle famiglie al cui interno ci sono soggetti che presentano la patologia della SMA (atrofia muscolare spinale) che necessitano appunto di ADI. soggetti che non deambulano, come nel caso del piccolo Christian di nove anni, che ha diritto a sessantacinque ore di assistenza infermieristica settimanale e che si serve di una struttura a cui l'ASL dà ben 13.000 euro mensili. Sono collegati a un ventilatore polmonare H24, necessitano di aspirazione salivare e hanno bisogno di essere aiutati con manovre e macchinari per espellere il catarro in abbondanza. Tuttavia questi soggetti, che avrebbero bisogno invece di vivere una vita piena,

Spesso questo personale viene formato nel corso degli anni per quel tipo di intervento specifico e poi viene reclutato da altri enti ospedalieri, spezzando inesorabilmente quel filo di relazione fiduciaria e affettiva che li lega al paziente. Nell'epoca del rilancio all'inclusione trovo che sia una pecca sociale, un *vulnus* di sistema enorme, consentire che questa problematica affligga ancora un numero di famiglie così esteso, peraltro già fragile e flagellato dal problema medico in sé. Per tutta questa serie di motivi sarebbe opportuno regolamentare le cure domiciliari con una disciplina adeguata e promuovere nelle sedi opportune dei progetti di assistenza personalizzata che prevedano la reintegrazione del personale formato per quel tipo di intervento. Il personale dovrebbe essere assunto dalle ASL o dalle Regioni con contratto a tempo indeterminato. Questa sarebbe una garanzia per le famiglie, perché in questo modo il personale non lascerebbe i pazienti per un incarico migliore, come accaduto nel corso degli anni. Le infermiere durante le ore di assistenza dovrebbero poter seguire il soggetto e, in special modo, il paziente, il bambino, ovunque lui voglia e debba andare - a scuola, alle visite mediche o a fare passeggiate - riducendo per le famiglie sensibilmente ulteriori costi in termini di altri assistenti o di proprie ore lavorative sottratte. Il progetto dovrebbe prevedere, oltre al personale infermieristico, anche figure quali fisioterapisti, logopedisti, anestesisti, cardiologi e assistenti specializzati. Vi ringrazio per l'intervento e spero che tutto ciò possa avvenire nel più breve tempo possibile. Ciao Christian.